*(PdL)*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nonostante la copiosa produzione legislativa del nostro Parlamento in materia di tutela dei minori, sono ancora tanti i nodi irrisolti nel panorama della responsabilità genitoriale, soprattutto quelli legati alle dinamiche del riconoscimento giuridico della stessa. Il nostro Paese in questi anni, ha man mano adottato tutta una serie di provvedimenti, misure e norme per adeguare al meglio le azioni ad un contesto sociale in continua evoluzione e in movimento da ogni punto di vista e di certo proprio ora non può correre il rischio di rimanere indietro rispetto agli altri Paesi europei, lasciando in sospeso situazioni inerenti a bambini sottratti, abbandonati, abbandonati, in difficoltà familiari, bambini che provengono da Paesi colpiti da calamità naturali o da Paesi in guerra e che hanno estremamente bisogno del nostro aiuto. A questo proposito, il 19 ottobre 1996, nell'ambito della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato, è stata redatta una convenzione riguardante la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Si tratta di una convenzione importante che contiene fondamentali provvedimenti di protezione internazionale dei minori adottati all'estero, che integrano quelle relative a materie già regolamentate, come l'adozione internazionale, la sottrazione dei minori, gli obblighi alimentari. alimentari. Attraverso la ratifica, infatti, gli Stati membri si impegnano: a dare il proprio contributo per creare uno spazio comune giudiziario e a costituire vie di comunicazione tra le autorità dei Paesi di origine e quelli di destinazione dei minori adottati; adottati; a determinare quale Stato sia competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore e la competenza delle autorità del Paese in cui il minore si trova fisicamente per l'adozione di tutti i provvedimenti di urgenza; di urgenza; ad individuare la legge applicabile dalle autorità competenti e la legge applicabile alla responsabilità genitoriale e, infine, a garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti e a stabilire una cooperazione tra gli Stati coinvolti nell'emanazione e nel riconoscimento minori. Come ricordavo, l'Italia, già firmataria di molti altri trattati internazionali in materia d'infanzia e dei suoi diritti, ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 1996 nel maggio del 2003, ma non ha ancora proceduto alla ratifica che è di fatto urgente anche in seguito alla decisione del Consiglio europeo del 5 giugno 2008 con cui l'Italia, fra gli altri Stati, è stata autorizzata alla ratifica stessa entro il 5 giugno 2010. È trascorso più di un anno da quella data e siamo certi che la ratifica della Convenzione sia ormai vicina. Come si sa, quando si gioca una partita secondo le regole fissate

è emerso che la principale difficoltà nel processo di ratifica discenderebbe dal riconoscimento dell'istituto della *kafala* previsto nella Convenzione. Negli ordinamenti musulmani la *kafala* è un istituto che consente di adempiere al dovere di fratellanza e di solidarietà nei confronti dei minori soli, orfani o abbandonati. In pratica due coniugi, o anche un singolo affidatario (il cosiddetto *kafil*), accolgono un bambino (*makful*) e si impegnano a nutrirlo, mantenerlo ed educarlo come fosse il proprio figlio. L'affidamento si protrae fino al compimento della maggiore età, ma non dà diritto all'eredità né all'acquisizione del nome del nucleo in cui il bambino viene inserito. In seguito ad un attento approfondimento sulla questione della e in concordanza con l'orientamento della Cassazione, si è giunti ad affermare che questo istituto sia conforme ai princìpi del nostro ordinamento nel caso in cui l'affidamento avvenga in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria locale (la cosiddetta *kafala* giudiziale) e non in base ad un semplice accordo di diritto privato tra le parti, anch'esso previsto dall'ordinamento islamico (*kafala* consensuale). Quest'ultima, infatti, consiste in un negozio giuridico che consente di cedere a un terzo le prerogative del genitore e presenta quindi l'evidente rischio di dissimulare forme di sfruttamento e schiavitù. orientamento condivisibile, che consente di collocare in Italia, entro parametri normativamente corretti, un istituto islamico riconosciuto dalle convenzioni internazionali. Proprio su questa delicata e importante questione si è espresso il comitato per l'Islam italiano presieduto dal ministro dell'interno Maroni che, tra l'altro, ha evidenziato come sia fondamentale che nella legge di recepimento di questo istituto sia garantita ai minori che vengono affidati ad adulti residenti in Italia la medesima tutela di cui godono gli altri minori, in particolare demandando al tribunale per i minori il il compito di accordare l'assenso e di esercitare i medesimi controlli previsti in caso di adozione internazionale. In ogni caso, per approfondire le modalità con cui procedere alla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione dell'Aja è stato costituito un tavolo interministeriale coordinato dal Ministero della giustizia a cui partecipano, tra gli altri, i rappresentanti del Ministero degli esteri, dell'interno, del lavoro, della salute e delle pari opportunità, che ha lavorato ad un testo che, avendo ancora bisogno di modifiche e perfezionamenti, non è ancora stato portato all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.

la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, firmata dal nostro Paese nel maggio 2003, non è stata ancora ratificata. La ratifica della Convenzione sarebbe dovuta avvenire entro il 5 giugno del 2010. L'Italia, quindi, non avendo ancora provveduto alla ratifica di tale Convenzione è sotto esame da parte dell'Unione europea e corre il rischio che vengano attivate le procedure contro la violazione dei trattati previste dall'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La ratifica della Convenzione, che costituisce l'aggiornamento di quella del 1961, oggi vigente nel nostro Paese, contribuirebbe a potenziare le politiche di tutela dei minori, sviluppando una cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, e condizionando i provvedimenti stranieri in tema di misure di protezione della persona e dei beni del minore al rispetto di una procedura che preveda la consultazione da parte dell'autorità giudiziaria competente dello Stato di residenza del minore. Tutto ciò si evince dal combinato disposto di numerosi articoli proprio di tale Convenzione; Convenzione; essa assume quindi un'importanza strategica per quanto concerne la protezione dei minori nelle situazioni di custodia di tipo internazionale che coinvolgono i diversi Stati. Non dimentichiamo i numerosi contenziosi, sotto gli occhi sotto gli occhi di tutti, di quei coniugi che in fase di separazione oppure di divorzio e con cittadinanza in Stati diversi rapiscono i propri figli al coniuge che aveva avuto l'affidamento in uno degli Stati membri dell'Unione europea. Tali contenziosi, purtroppo, sono ancora aperti. Il ritardo accumulato dal nostro Paese deve essere ricondotto in modo particolare al problema relativo al riconoscimento formale, inserito nella Convenzione in questione, dell'istituto della *kafala*. Qui si fa riferimento articolo 3, punto *e)*, e all'articolo 33 proprio della Convenzione. Il Ministero dell'interno, infatti,

l'istituto di diritto islamico della *kafala* trae la sua origine dal Corano che non ammette che possano essere rescissi integralmente i legami tra il minore adottato e la sua famiglia di origine; nei Paesi islamici fatta eccezione per la Turchia, la Somalia ed il Libano, l'adozione è vietata, oppure non le viene riconosciuto alcun valore. Nei Paesi islamici l'adozione legittimante è espressamente vietata dal Corano, perché rescinde i legami tra il minore e la sua famiglia. Pertanto, l'unico strumento di protezione del minore abbandonato è proprio la *kafala*. *Kafala* significa che una persona adulta si prende l'impegno di nutrire, curare e mantenere il minore fino al raggiungimento della maggiore età, senza il vincolo della filiazione e nemmeno la rottura dei rapporti giuridici con la famiglia di origine. È necessario ricordare che l'istituto della *kafala*, che presenta dei tratti molto simili ad una sorta di affidamento illimitato o *sine die*, è espressamente richiamato nella Convenzione ONU del 1989. Il Ministero dell'interno, in conformità con un consolidato orientamento della Cassazione, è intervenuto di recente con atti formali in merito all'istituto della *kafala*, evidenziandone la conformità ai principi del nostro ordinamento giuridico solo nel caso in cui l'affidamento avvenga in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria locale (attraverso la *kafala* giudiziale), e non in base ad un semplice accordo di diritto privato tra le parti (quindi,

e si presenta come una sorta di affidamento extra-parentale di minori, non creando alcun legame parentale tra gli adottanti ed il minore. La *kafala* consensuale può essere assimilabile ad un affidamento a tempo illimitato; è un istituto che non è previsto nella normativa delle adozioni e che, pertanto, non collima con il nostro sistema giuridico, tant'è che il tribunale dei minori di Trento ha stabilito, con una sua sentenza del 5 marzo 2002, che la *kafala* non può in alcun modo essere equiparata ad un affidamento preadottivo e non può essere dichiarata efficace in Italia. Attualmente, non a caso, i genitori adottivi italiani non si vedono riconoscere il provvedimento nel nostro Paese. Non solo, ma ai genitori adottivi che usufruiscono della *kafala* consensuale per adottare minori provenienti dai Paesi islamici viene richiesto anche di dichiarare, proprio nell'atto notarile privato, seppur formalmente, la conversione all'Islam. In data 6 ottobre 2010, nel corso dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata relativa all'argomento presso la III Commissione permanente della Camera dei deputati, il Governo all'argomento, il Governo ha dichiarato che lo scioglimento della riserva precedentemente posta da parte del Ministero dell'interno con riferimento alla sola *kafala* giudiziale, permette che vengano ripresi i lavori della commissione interministeriale preposta proprio ad estendere il testo del disegno di legge di ratifica della Convenzione dell'Aja, della quale stiamo trattando. Noi chiediamo come Lega Nord che il Governo si impegni quindi ad attivare tutte le procedure necessarie al fine di adempiere in tempi brevi alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ma anche ad introdurre, secondo le indicazioni già formulate e presentate presentate ufficialmente dal Ministero dell'interno nel tavolo di lavoro che vede coinvolti i Ministeri interessati per il completamento del testo del disegno di legge governativo di ratifica della convenzione, una particolare disciplina in relazione al riconoscimento dell'istituto della *kafala*. Chiediamo questo proprio per tutte le informazioni che con chiarezza ho messo in evidenza nell'illustrazione della nostra mozione e per garantire che prevalga il diritto di educazione, oltre che il dovere di curare ed amare il minore adottato, da parte della famiglia adottante secondo i propri convincimenti culturali, senza che essa debba soggiacere a vincoli che ne mortifichino o ne condizionino anche la libertà religiosa. Tutto ciò, a salvaguardia della nostra cultura, fondata anche sulla libertà di scelta educativa da parte di ogni singola famiglia, sulla libera assunzione di responsabilità verso i doveri della genitorialità, oltre che sulla grande generosità delle famiglie italiane che decidono e ottengono di adottare minori.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, che questo Governo e questo Parlamento siano sensibili e siano impegnati

alla Convenzione sui diritti del fanciullo attraverso l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Purtuttavia dobbiamo riconoscere che da più di un anno è scaduto il termine fissato dal Consiglio dell'Unione europea per la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996. della Convenzione dell'Aja del 1996. Tale Convenzione, che riguarda la responsabilità genitoriale e la protezione dei minori, è sicuramente da considerare un valido strumento per il miglioramento della cooperazione tra Stati in materia di protezione dell'infanzia. Infatti, la sua applicazione consentirebbe sicuramente di dare tante risposte e di adottare tutti quei provvedimenti su migliaia di bambini e di adolescenti che si trovano in difficoltà. Mi riferisco ai cosiddetti bambini non accompagnati che provengono dai Paesi del Nord Africa, bambini sicuramente in difficoltà familiari, bambini provenienti da aree sede di conflitti militari o colpiti da catastrofi naturali.

applicazione risolverebbe e supererebbe tutte quelle problematiche che diventano situazioni limite dal punto di vista giuridico perché i sistemi giuridici non collaborano tra di loro, non dialogano tra di loro. Tra questi abbiamo il riconoscimento della *kafala*, come ampiamente descritto nelle varie mozioni, varie mozioni, un istituto che non è riconosciuto ancora dallo Stato italiano e che quindi non permette ai minori abbandonati provenienti dal Nord Africa di essere accolti dalle aspiranti famiglie adottive residenti in Italia. Eppure sappiamo che sono tantissimi i bambini abbandonati nel Nord Africa: solo nel Marocco ne abbiamo circa 60.000. Si tratta di bambini neonati abbandonati e bambini di strada, che vivono nei centri senza aver alcun legame con la famiglia o con i familiari in genere. genere. Questi minori, pur essendo abbandonati a loro stessi, non possono essere affidati perché l'Italia non riconosce questo sistema di protezione dell'infanzia che è la *kafala*. La Convenzione dell'Aja del 1996 prevede proprio questo tipo di consultazione tra varie autorità del Paese di origine del minore e del Paese di residenza, per garantire l'accoglienza familiare. familiare. L'augurio è che al più presto il Governo possa accogliere e ratificare questa Convenzione perché in questa maniera

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, nel 1996 si è provveduto alla firma e alla relativa ratifica, da parte degli Stati membri, della Convenzione dell'Aja concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori a livello internazionale, che integrano quelli già regolamentati dai singoli Stati. Da allora, in materia di responsabilità genitoriale, sono stati adottati o proposti numerosi atti, in particolare il regolamento (CE) n. che aveva previsto il riconoscimento reciproco di certe decisioni in materia di responsabilità genitoriale emesse in occasione di un divorzio o di una separazione

impegnando gli Stati membri a creare uno spazio giudiziario comune. Essa, infatti, è applicabile ai provvedimenti che riguardano bambini e adolescenti ostaggi di sistemi giuridici nazionali che non dialogano fra loro (minori provenienti da Paesi colpiti da calamità naturali, minori in affido internazionale, minori con provvedimento di *kafala*). L'esempio più eclatante riguarda il riconoscimento della *kafala*, la più alta forma di protezione dell'infanzia abbandonata nei Paesi dell'Islam, ed è proprio questo il punto critico nel processo di ratifica. Germania, Francia, Irlanda e Regno Unito nell'anno 2010 hanno provveduto a ratificare la Convenzione dell'Aja, mentre invece non c'è ancora nessun segnale dall'Italia, unico tra i grandi Paesi della Comunità europea a non aver ancora dato una risposta chiara alle sollecitazioni delle istituzioni europee rispetto alla ratifica di una Convenzione definita dallo stesso Consiglio dell'Unione europea «di rilevanza comunitaria». scaduto - com'è stato detto in quest'Aula - il 5 giugno dell'anno scorso il termine fissato dal Consiglio dell'Unione europea per la ratifica del testo della Convenzione del 1996 da parte dell'Italia e di altri Paesi Sappiamo che il tavolo interministeriale coordinato dal Ministero della giustizia a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro, della salute e delle pari opportunità sta procedendo con impegno ai lavori, ma è proprio per questo che dobbiamo provvedere alla presentazione di una norma in tempi molto brevi che autorizzi la ratifica della Convenzione dell'Aja.

ha voluto valutare scrupolosamente tutte le disposizioni destinate a trovare applicazione nel diritto nazionale.

*(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, signora Sottosegretario, come ho già avuto modo di dire in sede di illustrazione, credo che i tempi siano maturi per procedere finalmente alla presentazione dell'apposito disegno di legge di ratifica della Convenzione dell'Aja sui minori. Vorrei tuttavia precisare ancora una volta che il fatto che il termine per la ratifica della Convenzione fosse preferibilmente fissato al 5 giugno 2010 non autorizzava nessuno a lasciarlo spirare con tanta leggerezza.

Il dibattito ha comunque dimostrato che la ratifica

darà oggi un altro segnale forte di sensibilità sui temi dell'infanzia, dopo la recente e condivisa approvazione della legge sull'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia. Tuttavia restano aperte alcune serie e concrete problematiche. Per quanto riguarda le risorse, persiste il problema della mancanza di bilanci che rendano trasparenti le risorse dedicate all'infanzia e all'adolescenza in Italia. La legge di stabilità del 2011 ha diminuito i fondi della legge n. 285 del 1997 e lo stesso fondo è stato poi diminuito di un altro 10 Per quanto riguarda la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, va rilevato che dal 2010 vi è un cambiamento nel metodo di conteggio. Fino al 2010 la quota del fondo considerava gli oneri obbligatori per i diritti soggettivi (agevolazioni a genitori di bambini con disabilità, assegni di maternità, assegni ai nuclei familiari, indennità per i lavoratori affetti da talassemia *major*) più i fondi destinati alle Regioni, alle Province autonome e la quota imputata al Ministero per il suo funzionamento istituzionale. Dal 2010 la quota del fondo si deve calcolare al netto degli oneri per i diritti soggettivi. Abbiamo assistito negli anni ad una netta diminuzione del fondo; questa situazione è stata sottolineata anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ha espresso la propria preoccupazione per i tagli al fondo nazionale per le politiche sociali,

Sono stati drasticamente ridotti i Fondi per le politiche della famiglia (da 186,6 milioni di euro nel 2009 a 51,475 milioni di euro del 2011), per le pari opportunità (da 40 milioni di euro nel 2009 ai 17,256 milioni di euro per quest'anno) e del Fondo per le politiche giovanili (da 79 milioni di euro a 12,788 milioni di euro per il 2011). Questi fondi non riguardano direttamente l'infanzia e l'adolescenza, ma hanno ovviamente un impatto sui minori in Italia. Nel 2011 sono rimasti invariati i fondi destinati all'infanzia nel quadro della cooperazione internazionale, ma i fondi complessivamente destinati alla cooperazione diminuiscono. La legge di stabilità ha infatti tagliato del 46 per cento i finanziamenti alla cooperazione e dal 2008 gli stanziamenti per la legge n. 49 del 1987 sono scesi del 78 Ricordo infine che il Piano nazionale per l'infanzia è stato approvato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 9 maggio scorso. Prima della sua approvazione, il Piano era stato esaminato dalla Commissione bicamerale infanzia e dalla Conferenza Stato-Regioni. La Commissione bicamerale, dopo un'indagine conoscitiva, iniziata il 5 ottobre 2010 e conclusa il 28 ottobre 2010, nel febbraio 2011 aveva dato parere favorevole al Piano, pur evidenziandone alcuni aspetti critici. Si è espressa invece in senso sfavorevole sullo schema del Piano nazionale la Conferenza Stato-Regioni. Ma ciò che è più preoccupante è anche in questo caso la mancanza di fondi *ad hoc* per l'attuazione del Piano. Signor Presidente, credo che affrontare queste questioni sia necessario e doveroso oggi ancor di più, mentre si approssima un ennesimo pesantissimo intervento in materia finanziaria. Si proceda all'approvazione di un'adeguata normativa a tutela dell'infanzia, ma si provveda anche a fornire gli strumenti adeguati perché questa normativa possa effettivamente trovare concreta applicazione. *(Applausi del

Signor Presidente, non mi soffermerò ulteriormente sull'importanza di questa Convenzione sostanzialmente mira a creare delle norme uniformi per individuare l'autorità nazionale competente a decidere in materia minorile, in modo da evitare provvedimenti contrastanti da parte di due Stati diversi. Voglio ancora dire che effettivamente c'è stato un ritardo da parte dell'Italia nella ratifica della Convenzione, ma la formula usata nel Consiglio dell'Unione europea del 5 giugno 2008 e, cioè, giungere alla ratifica «se possibile anteriormente al 5 giugno 2010» mi porterebbe ad escludere che lo sforamento di questo termine possa configurare un inadempimento italiano. Quindi, l'idea che in base a questo possa esserci una sanzione da parte dell'Europa, a mio avviso, non corrisponde al vero. Perché c'è stato questo ritardo? Forse si poteva fare più in fretta, ritengo però giusto lo studio che è stato fatto e credo che sia giusto riconoscere al Ministero dell'interno che si è espresso in conformità con un orientamento della Cassazione più volte formulato, secondo il quale con il nostro ordinamento è compatibile l'istituto della *kafala* solo nel caso in cui l'affidamento avvenga in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziale locale (appunto la *kafala* giudiziale) e non in base a un semplice accordo di diritto privato tra le parti, che anch'esso sarebbe compatibile con l'ordinamento islamico (la *kafala* consensuale), ma che consiste in un negozio giuridico che consente di cedere ad una terza parte le prerogative del genitore e presenta il rischio di dissimulare forme di sfruttamento e schiavitù; non è sicuramente questo che noi vogliamo. Questa è stata la preoccupazione anche di molti altri Stati, come il Belgio e la Germania, che hanno risolto anch'essi dando maggiore importanza alla *kafala* giudiziale ed escludendo altre forme di *kafala*. È questo uno sprone al Comitato interministeriale per arrivare al più presto all'approvazione della legge di ratifica che, ripeto, è e sarà un vantaggio

onorevoli colleghi, con l'approvazione delle mozioni che ci apprestiamo a votare, aggiungiamo un altro importante tassello all'impegno che in quest'Aula, in maniera costante negli ultimi mesi, abbiamo voluto manifestare e perseguire in tema di protezione dei minori e responsabilità genitoriale. La recente istituzione del Garante per l'infanzia ne è una prova, ma occorre anche ricordare la ratifica della Convenzione di Lanzarote in tema di violenza sui minori e pedofilia, il provvedimento sulla competenza in tema di potestà genitoriale che ha equiparato i figli naturali e legittimi davanti al tribunale ordinario, quello a favore dei figli di detenute madri e molti altri ancora. In generale, va poi ricordato come l'Italia abbia tentato, negli ultimi anni, di velocizzare l'accidentato percorso di ratifica delle Convenzioni dell'ONU ed europee, che hanno sempre richiesto, per loro natura, tempi lunghi e *iter* sofferti. È questo il caso anche della Convenzione dell'Aja del 1996, che ha trovato il principale ostacolo nella oggettiva difficoltà ad adeguare uno strumento previsto dal diritto islamico e sconosciuto al nostro ordinamento come la *kafala*, in quanto confliggente con altri istituti del nostro ordinamento apparentemente simili, ma in punto di diritto fortemente diseguali. Le difficoltà che il Governo italiano ha sin qui evidenziato scaturiscono da fondati dubbi circa la possibile strumentalizzazione e l'abuso della stessa *kafala*, ove non adeguatamente normata, Lo scopo di questa Convenzione è invece proprio quello di creare uno spazio comune giudiziario e quindi di ridurre i conflitti tra legislazioni, in particolare individuando la legge applicabile, il riconoscimento, 1'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e protezione dei minori. minori. Vogliamo dare atto al Governo del grande lavoro svolto in sede interministeriale e parimenti del grande apporto tecnico e culturale che il Comitato per l'Islam, insediato presso il Ministero dell'interno, ha voluto fornire alla vicenda. Dobbiamo inoltre darci conto del fatto che l'Italia, diciamolo con orgoglio, il nostro Paese, ha saputo anche nel passato più recente e nell'attualità essere in prima linea, in special modo nei confronti dei minori e degli adolescenti, per solidarietà, accoglienza e integrazione: ben oltre la disponibilità che ci aspettavamo, e non è arrivata, da quei Paesi a noi storicamente e culturalmente più vicini. Delle stime ci dicono che i minori non accompagnati, sbarcati a Lampedusa solo nel mese di maggio, sarebbero circa 500. Questa è la verità, una verità ancor più vera quando storie anonime diventano voci, volti, occhi di bambini e bambine che chiedono di vedersi riconoscere, in qualsiasi modo, il diritto primario di essere circondati di affetto, affetto e ancora affetto. Questo è bene ribadirlo: che si parli di *kafala*, o adozione o affido, al centro deve sempre essere l'interesse del minore, il suo sviluppo, la sua educazione, la sua crescita. Che si parli di *kafala*, o adozione o affido, nessuno può pensare di eludere il rispetto della legge. L'Italia, è bene ricordarlo, proprio per le verifiche e i controlli pre e post adozione, con una normativa rigorosa e protocolli altrettanto puntuali si è guadagnata un ruolo *leader* in materia nel mondo. Attorno a questo nodo ruotano interrogativi e dubbi sin qui avanzati dal Governo, al quale chiediamo di inviare presto alle Camere un testo equilibrato, una sintesi che, tenendo conto delle diversità culturali e religiose di una società multietnica, ribadisca i paletti normativi (è stato già ribadito il distinguo tra *kafala*

fare una riflessione complessiva: per esempio, la realizzazione della banca dati dei bambini adottabili, la riduzione del numero (16.000 circa) di minori che trascorrono l'intera infanzia e adolescenza in istituti a causa di rinnovi *sine die* dei decreti di affidamento, o anche 1'esclusione a tutt'oggi di ciò che invece la Convenzione dell'Aja del 1993 sulle adozioni consente, e cioè 1'adozione in uscita per quei minori adottabili che non trovano famiglia in Italia. Queste mozioni hanno oggi, simbolicamente, la faccia di Munir, il bambino egiziano affidato in *kafala* ad una famiglia italo-egiziana delle Marche e ancora in orfanotrofio per il rifiuto del visto. Ma la Convenzione dell'Aja del 1996 sui minori è molto di più: per esempio, un efficace strumento per combattere quel triste e crescente fenomeno dei minori non accompagnati in Italia che spesso rappresenta solo l'anticamera della loro scomparsa,

e lo accompagni verso la vita e che ne faccia prima un uomo o una donna e dopo un cittadino. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni. Metto ai voti la mozione n.

che impegnano il Governo a produrre gli atti per la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996 finalmente - e sottolineo finalmente - il Parlamento dimostra di voler mettere l'Italia al pari con gli altri Paesi in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Lo facciamo tuttavia con tanto ritardo rispetto a tutti gli altri Paesi dell'Unione; inoltre, considerando che questa Convenzione era stata sottoscritta dall'Italia nel maggio 2003, il nostro giudizio non può che essere articolato. Non possiamo sottacere infatti lo scandalo della mancata approvazione lo scorso anno e fin qui di questa che è forse la più importante Convenzione recente per la protezione dei minori. Già da molto tempo la ratifica avrebbe consentito all'Italia di sbrogliare quella vera e propria intricata matassa che tuttora impedisce a migliaia di minori abbandonati di essere accolti da famiglie italiane. Infatti, questa Convenzione troverebbe applicazione per tutti quei provvedimenti che interessano bambini e adolescenti in ostaggio di sistemi giuridici nazionali che non sono capaci di dialogare tra loro. L'esempio più clamoroso è forse quello del mancato riconoscimento della *kafala*, di cui tanto abbiamo parlato, ovvero di quello che è considerato il più alto e diffuso strumento di protezione dell'infanzia negli Stati nordafricani. L'Italia, a differenza di altri Paesi europei, si è troppo a lungo attardata nel mancato riconoscimento di questo istituto senza peraltro saper individuare fino ad ora strade e soluzioni sostenibili e percorribili per dare possibilità concrete e legali ai minori abbandonati di essere accolti da una famiglia italiana. Pensiamo ad esempio che in Marocco sono più di 60.000 i minori abbandonati che vivono senza una famiglia. Il caso del Marocco si distingue dagli altri proprio perché nella maggioranza dei casi questi minori non hanno legami con le famiglie di origine,

origine, ma non possono essere accolti in Italia perché il nostro Paese non ha riconosciuto la *kafala* come sistema di protezione dell'infanzia. Ecco, la Convenzione dell'Aja del 1996 è stata pensata e voluta proprio per questo motivo, per superare questa *impasse* giuridica, prevedendo procedure di consultazione tra le autorità di due Paesi per garantire l'accoglienza di minori presso le famiglie. Così come la Convenzione dell'Aja del 1993 ha contribuito a regolamentare il sistema dell'adozione internazionale garantendo trasparenza e rigore alle politiche per l'accoglienza familiare di 81 Paesi del mondo, così l'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1996 permetterà di dare risposta a migliaia di casi di minori abbandonati o di fatto oggetto di veri e propri ostracismi burocratici. Dei diritti dei bambini si parla certamente molto, ma troppo spesso si perdono di vista le vie più semplici, quelle più adatte a tutelarli. E dobbiamo sapere che tutte le azioni o le omissioni che rallentano la possibilità di accogliere un bambino un bambino costituiscono, di fatto, azioni concrete contro quel bambino o bambina. La mancata ratifica fino ad ora ha certamente messo in luce un disinteresse del legislatore e della maggioranza di Governo, ma forse anche l'intento di qualcuno di contrastare i principi stessi di quella Convenzione. Si tratta di ritardi, inerzie, dilazioni che il nostro Paese sta pagando duramente, a prezzo della sua stessa considerazione nel nel consesso internazionale ed europeo. Sono troppi i casi di Trattati sottoscritti e non ratificati, ed esiste il rischio concreto, anche in questo caso, dell'attivazione di quelle procedure previste dalla Commissione contro la violazione dei Trattati: procedure gravissime per il nostro Paese, sia sotto il profilo della giurisdizione dinanzi alla Corte di giustizia sia per le sanzioni economiche previste. Tuttavia il voto unitario su queste mozioni mozioni ci fa ben sperare. E desidero veramente ringraziare tutte le senatrici, molte, e i senatori, pochi, di maggioranza e di opposizione, che si sono impegnati per questo importante risultato; e per il mio Gruppo, il Gruppo del Partito Democratico, desidero ringraziare in particolare la senatrice Anna Maria Serafini, che da anni, con decisione e grande competenza, si batte per garantire in pratica i diritti dei minori e degli adolescenti. Concludo con le parole de «Il Profeta», un «I vostri figli non sono vostri. Sono figli e figlie della vita che solo di se stessa ha desiderio. Ne siete lo strumento e non l'origine.... Vi potete sforzare di essere come loro, ma non pensare di farli come voi». Parole alte, universali, che suggeriscono di aprirci all'altro come misura e necessità di una vita civile.

che tutte le mozioni presentate contengono elementi e spunti di grande interesse, a testimonianza che il problema del gioco d'azzardo ha tante sfaccettature. È un fenomeno proteiforme, complesso e per certi aspetti ancora inesplorato. Voglio anche sottolineare in premessa che questo, a mio giudizio, deve essere l'avvio di un dibattito su questo tema. Non può essere in questa legislatura la conclusione, in quanto la Commissione parlamentare antimafia

la Commissione antimafia, tra pochi giorni, approverà un secondo rapporto, molto più articolato e dettagliato....

Il Comitato antiriciclaggio dell'Antimafia, dopo alcuni mesi di lavoro, sotto la presidenza del senatore Li Gotti, e dopo decine di audizioni che hanno visto presenti in Comitato tutti i settori investiti direttamente o indirettamente da questo problema, sottoporrà come proposta alla Commissione plenaria un documento che sarà inviato alle Camere per un dibattito approfondito. Quindi, questo è l'avvio di un dibattito e non la conclusione. Tuttavia serve per misurare l'urgenza dei problemi intorno alla questione gioco d'azzardo e l'esigenza di pervenire all'approvazione di misure urgenti sulla tutela dei minori, sul divieto di pubblicità ingannevole, sul controllo delle scommesse e dei percorsi finanziari intorno alle scommesse, sull'interdizione del riciclaggio del denaro sporco nelle scommesse e anche, cosa più interessante, per avere finalmente la trasparenza assoluta di tutti i concessionari di gioco. E allora, solo allora sarà possibile fare un'analisi globale di questo fenomeno e porsi degli interrogativi fondamentali:

si sottraggano risorse al gioco clandestino e quindi al dominio su di esso della criminalità organizzata; se risulta vero che, espandendo all'infinito il mercato del gioco, si ha un progresso dell'innovazione tecnologica, come qualcuno ha testimoniato nel Comitato antiriciclaggio; se espandendo all'infinito il mercato del gioco, ne deriva un aumento delle entrate erariali (questo non è un punto secondario); se esiste una reale discontinuità tra il gioco d'azzardo cosiddetto lecito e il gioco d'azzardo illecito, clandestino e controllato dalla criminalità organizzata. Se dovessimo fare riferimento alle molte indagini alle molte indagini in corso da parte della magistratura inquirente e delle forze di polizia, dovremmo dire che nei territori a sovranità criminale questa discontinuità non esiste, perché spesso i titolari delle agenzie sono prestanome, sono teste di legno della rete criminale. Allora, dovremmo rispondere a tutte queste domande, ma anche ad un'altra domanda, se l'attuale assetto amministrativo dell'AAMS, cioè dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al di là dei meriti dell'attuale dirigenza,

del sistema sanzionatorio e del sistema di verifica, consenta di tenere sotto controllo e in parte di arginare la dimensione crescente di questo fenomeno. Ripeto, è una domanda E non è colpa di nessuno se la rapidità espansiva di questo mercato ha costretto il Governo e il Parlamento a varare progressivamente progressivamente delle misure di adeguamento, ma che risultano sempre in ritardo rispetto alla dimensione globale del fenomeno. Ecco perché

nella mozione n. 202 (testo 2) ci sono alcune richieste al Governo - convergenti con altre richieste di altre mozioni - che riguardano, in attesa di questo documento dell'Antimafia e di una più approfondita analisi nelle sedi parlamentari e governative, la necessità di varare misure urgenti.

ad attivarsi per prevenire e reprimere il gioco d'azzardo illegale e le interazioni con il reticolato della criminalità organizzata mafiosa; ad intervenire con misure urgenti al fine di regolare in modo maggiormente rigoroso il gioco legale, ampliando le misure già previste nel Patto di stabilità; ad individuare gli strumenti più idonei alla trasparenza delle licenze; ad adottare misure di controllo sui giochi telematici; ad introdurre più stringenti norme a tutela dei minori. Le richieste di questa mozione vanno proprio nella direzione delle misure urgenti di cui parlavo prima. Presidente, colleghi, anch'io illustrerò brevemente la mozione n. 222. Il gioco d'azzardo affonda le radici nella storia antica e coinvolge sempre più cittadini, pensionati, fasce deboli, accomunati dalla speranza di avere fortuna e di cambiare la propria vita. Il fenomeno diventa patologico; c'è una dipendenza da gioco che coinvolge sempre più cittadini e assume dimensioni di una vera e propria emergenza sociale. Un recente rapporto dell'Eurispes, fotografando la situazione italiana, ha evidenziato che le persone patologicamente dipendenti dal gioco legale e d'azzardo sono stimate in circa 700.000 unità, delle quali circa l'85 per cento sono uomini.

Il fenomeno risulta anche diffuso tra i giovani, molti dei quali impegnano in tali attività somme di denaro ragguardevoli in rapporto all'età e alle risorse disponibili, soprattutto nel Meridione, dove un'incidenza dei giochi rispetto al reddito *pro capite* molto elevata; addirittura in provincia di Caserta viene utilizzato per le giocate il 12,7 per cento del reddito *pro capite*. Molte associazioni a scopo non lucrativo sono nate per tamponare l'emergenza sociale. Tuttavia, al di là dei numerosi sforzi, l'ampiezza del fenomeno è tale da richiedere un urgente intervento da parte dello Stato e del Governo. L'azzardo è divenuto progressivamente un bene di consumo promosso come occasione di scambio sociale, con promesse di vincite facili e cospicue. I giochi d'azzardo non creano abilità bensì distruggono sogni e vite. Ci rendiamo conto che è difficile rinunciare a 65-70 miliardi di euro l'anno (a tanto è arrivato il giro di affari però se Federalberghi-Confturismo ha lanciato l'allarme di un aumento inevitabile di meccanismi pericolosi che già girano intorno ad alcune case da gioco, al cui interno si innestano fenomeni criminali, come l'usura e l'estorsione, lo Stato si deve porre questo problema. In Italia ci sono 800.000 nuovi disoccupati tentati dal ricorso alla fortuna attraverso la continua proposta di giochi, che finisce per affamare ulteriormente le persone più deboli. Incentivare il gioco d'azzardo vuol dire aumentare quelle vittime di cui poco si tiene conto, i giocatori patologici. Essi sono seguiti e curati quasi esclusivamente da associazioni di volontariato; nascono le cliniche per la disintossicazione. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 152 del 1985, denunciando la necessità di una legislazione organica che razionalizzasse il settore, auspicando una revisione dell'attuale disciplina.

tende soprattutto a denunciare il ruolo svolto dalla criminalità organizzata, che si è infiltrata e che gestisce una quota rilevante del mercato. Dalla metà degli anni Ottanta, i casinò italiani hanno subito delle operazioni strutturate della criminalità organizzata volte a controllare i flussi legali del gioco d'azzardo e l'indotto. Il connubio tra giochi pubblici e giochi clandestini è divenuto ormai una drammatica realtà. La nostra mozione quindi impegna il Governo ad attivarsi al fine di evitare che le famiglie italiane, attratte dal miraggio del facile e immediato arricchimento, in una situazione di massima crisi economica accompagnata da pesante disoccupazione, continuino a precipitare in vere e proprie forme di dipendenza patologica da gioco; ad adottare forme di tutela degli utenti del gioco *online* al fine di evitare abusi, specialmente per quanto concerne i giochi di carte; ad adottare iniziative finalizzate ad evitare che la criminalità organizzata continui a trarre il massimo profitto dal settore dei giochi e delle scommesse; a ridisegnare l'intera disciplina del settore del gioco al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e alla diffusione del gioco irregolare, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, ed assicurare, altresì, la tutela del giocatore; a destinare, infine, parte dei proventi derivanti dalla raccolta conseguente ai giochi e alle scommesse ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla definizione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Concludo, signor Presidente, confidando nell'accoglimento

i più deboli, le fasce più deboli cercano nel gioco di migliorare le proprie condizioni di vita.

Signor Presidente, il gioco d'azzardo credo possa essere definito un'urgenza nell'agenda politica e uno dei mali che indebolisce e impoverisce, sicuramente dal punto di vista materiale ma anche morale e - oserei dire - antropologico, la nostra società. L'Istituto superiore di sanità definisce la patologia del gioco d'azzardo come una dipendenza, sicuramente un dipendenza senza sostanza: potremmo parlare di ludodipendenza.

delle forze politiche che siedono qui in Senato, ricordando che l'articolo 721 del codice penale definisce giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. È proprio su questa vincita aleatoria che si muove il motore dell'industria dei giochi, che in fondo è la terza industria italiana, preceduta solo da ENI e da FIAT. Parliamo di un giro di denaro da capogiro: è un gioco di parole, ma ritengo che permetta di spiegare quello di cui stiamo parlando parlando oggi. Nel 2010, infatti, gli italiani hanno speso, per giochi di azzardo e scommesse, più di 61 miliardi di euro, con un incremento del 13 per cento rispetto all'anno precedente, e per il 2011 si stima che la spesa raggiungerà gli 80 miliardi di euro. Con Internet sono proliferati i giochi *on line*, tanto che, secondo una nota dei Monopoli di Stato, nel 2010 le relative entrate sono cresciute del 28,2 per cento rispetto all'anno precedente. Tutto questo vuol dire che, di fatto, oggi circa l'80 per cento della popolazione adulta gioca d'azzardo. Quel che peggio è che maggiormente dediti al gioco sono proprio le persone più deboli,

Proprio guardando queste cifre si avverte la gravità del fenomeno. È stato stimato che, in Italia, circa 700.000 persone, il 3 per cento dei giocatori, sono vittime del gioco patologico e che 7 milioni di persone, il 26 per cento dei giocatori, sono considerati dei soggetti a rischio. Parliamo di persone che hanno stabilito con il gioco di azzardo una vera e propria relazione di dipendenza. Tali percentuali sono destinate a crescere.

Si legge che si vuole introdurre nei supermercati la possibilità di giocare: i clienti, sostanzialmente, per arrotondare il costo della spesa alimentare, potranno rischiare al massimo fino a cinque euro, scegliendo di trasformare il resto della spesa in una ricevuta di partecipazione a una estrazione a premi. Questo è allarmante, se consideriamo che quei dati sono dei dati oggettivi: non sono frutto di supposizioni, ma sono dati riportati anche nei documenti e nelle relazioni che il Governo presenta al Parlamento. Quello di cui si parla nell'articolo 721 del codice penale, quindi, questo sogno aleatorio, è un sogno che ci deve preoccupare. Speriamo che il Governo non attui questa scelta per raccogliere delle risorse. È una sorta di induzione in tentazione, e credo che sia terribilmente sbagliata. Ieri è stata presentata al Parlamento la relazione annuale sull'uso delle sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia. Parlando di dipendenze, è stato indicato proprio il gioco di azzardo come una fonte di rischio tale che, in particolare per i gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza. Nella relazione si sottolinea come i fenomeni di *gambling* patologico non siano stati inseriti nei LEA: lo si dice nella relazione del Governo. Per questo motivo, è difficile organizzare forme di cura e riabilitazione attraverso l'attuale sistema sanitario regionale. Vorrei ricordare che in Italia esistono 186 centri pubblici che si occupano già del gioco di azzardo patologico, e lo Stato, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, ha l'obbligo di garantire uniformità di tutela su tutto il territorio nazionale e di promuovere una politica di prevenzione e formazione. Sempre nella relazione annuale, si segnala che in Italia, sulla popolazione generale, i dati indicano una prevalenza di *gambling* patologico nel corso della vita pari all'1 per cento della popolazione appare a rischio di sviluppo della patologia. Nella popolazione studentesca, purtroppo, questa percentuale aumenta: è pari al 10 per cento. Secondo un'indagine della società

Dal punto di vista sociale i soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico rischiano di compromettere la loro vita finanziaria e la loro vita personale e, conseguentemente, la distruzione di legami familiari e lavorativi, fino ad arrivare alla richiesta di prestiti usurari: tra il 2005 e il 2010, infatti, si è osservato un aumento del 165

anche il suicidio. Se il Governo fosse davvero interessato a risolvere questo problema - e sono certa che il Governo risponderà da questo punto di vista cercherebbe di inserire nei livelli essenziali di assistenza la patologia del gioco d'azzardo. Nei primi cinque mesi del 2011, la Guardia di finanza ha annunciato di aver chiuso oltre 800 punti non autorizzati alla raccolta scommesse, ma almeno altrettanti ne sono stati aperti. Non solo. La passata legge di stabilità ha previsto che nel corso di quest'anno saranno immesse nel mercato 54.000 *slot machine*, oltre ai 300.000 apparecchi già esistenti. Di fronte a questa allarmante fotografia, è significativo che oggi il Senato abbia scelto di discutere queste mozioni. È un atto di grande responsabilità: le mozioni sono diverse ma sono complementari, ad affrontare la degenerazione che il gioco d'azzardo sta manifestando fortemente nel nostro Paese. Serve che lo Stato lanci un messaggio chiaro ed inequivocabile: ed inequivocabile: puoi giocare ma non puoi affidarti alla dea bendata per costruire un futuro migliore per te e per la tua famiglia. Insieme dobbiamo porre fine a queste scelte contraddittorie.

si dice che tutte le politiche devono essere analizzate anche dal punto di vista sanitario: speriamo che non vengano poi introdotti degli incrementi ai giochi d'azzardo. Non si tratta di dire no

Il nostro Stato democratico non può pensare di risanare i nostri conti pensando di attingere solo ai fondi derivanti dal gioco d'azzardo. Quindi, nella mozione chiediamo al Governo di impegnarsi ad inserire nei LEA i disturbi e le complicanze che si diagnosticano come conseguenza del gioco d'azzardo patologico, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la presa in carico delle persone affette da ludopatia e di individuare un percorso terapeutico, in modo che tutti coloro che sono affetti da gioco d'azzardo patologico non si sentano soli. Il Governo deve impegnarsi ad adottare gli opportuni atti di competenza per promuovere un programma di prevenzione e formazione e deve anche estendere - io chiedo - il gratuito patrocinio a spese dello Stato a favore dei soggetti affetti da ludopatie. Le loro famiglie rischiano davvero di cadere in una condizione di povertà. Purtroppo, essendomi occupata di questo argomento, sono venuta a conoscenza di situazioni davvero difficili. Vorrei concludere citando le parole del celebre poeta e filosofo libanese Gibran, il quale dice: «Il valore del vostro Governo non va ricercato in ciò che avete fatto, ma in ciò che avreste dovuto fare». Speriamo di farlo Confido, quindi, nel buon senso e nel senso morale di tutta l'Aula e del Governo affinché si possano muovere i primi passi di un progetto politico condiviso volto alla cura e alla prevenzione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico. Anche le altre mozioni affrontano questo aspetto, e mi auguro che ci sia un'approvazione corale. È un messaggio positivo quello che stiamo lanciando, perché con l'approvazione di queste mozioni diciamo chiaramente che non ci si può affidare al fato per «vincere» i momenti di debolezza e di difficoltà che possono attanagliare la nostra vita. Oggi vogliamo iniziare a vincere uno dei più grandi mali della nostra società e cercare di dare speranza alle persone che ne sono affette.

Non possiamo però non guardare in faccia la realtà e non accorgerci del fatto che stanno proliferando una serie di giochi. Il momento di crisi che si sta attraversando non fa che acuire posizioni di debolezza in grandi strati sociali, e il tentativo di risolvere i problemi con il colpo di fortuna - questo lo possiamo vedere - è sempre più frequente. Se andiamo a verificare i dati sulla diffusione dei videogiochi d'azzardo, sembra che in Italia si spendano 60 miliardi euro Se consideriamo che la popolazione italiana è pari a circa 60 milioni di persone, vuol dire che in media ogni cittadino spende in giochi più di 1.000

Cosa accade in determinati settori quando si è voluto frenare un certo tipo d'abitudine? Parlo del fumo e di quello tra i minori. tra i minori. Al di là della proibizione di vendere sigarette ai minori, si è trovato l'*escamotage*, stante che il sistema del distributore automatico è sempre più di un sistema per impedire ai minori di estrarre dalle macchiette automatiche i pacchetti di sigarette. Lo si è fatto con un sistema relativamente semplice: si deve introdurre la tessera sanitaria la quale, avendo riportati

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, l'industria dei giochi e delle scommesse è in continua e fortissima crescita con una raccolta che ha raggiunto nel 2010 i 61 miliardi e mezzo di euro con un incremento di più di 7 miliardi rispetto al 2009, generando anche un grosso introito per le casse dell'erario. Questo *trend* sta proseguendo in progressione geometrica. Nei primi sei mesi del 2011 la raccolta dei giochi pubblici ha superato i 36 miliardi, con un dato in crescita del 20 per cento rispetto

La fetta più consistente in termini di incassi arriva dalle *new* *slot* e dalle *videolottery*, che valgono oltre il 56 per cento del mercato complessivo; ma - se mi si passa l'espressione - tirano anche il gratta e vinci (15 per cento del totale) e il lotto (10 per cento). Infine, la previsione di raccolta complessiva del gioco *on* *line* viene stimato che possa raggiungere, per l'anno in corso, gli 11 miliardi Dunque c'è stata una crescita tumultuosa. Credo che si debba riconoscere che nell'arco degli anni si è operato intelligentemente per prosciugare un terreno di coltura del gioco illegale e di opacità, trasferendolo il più possibile nell'ambito del anche se, agendo di rincorsa e pressati dalla ricerca di massimizzazione degli introiti per l'erario, non sempre si è proceduto con appropriatezza. Troppe novità introdotte per decreti-legge, qualche elasticità nell'applicazione delle norme, scadenze via via spostate, decisioni poi corrette e rivisitate, controlli e sanzioni non sempre stringenti come necessario. Le audizioni della Commissione antimafia - lo ricordava il collega senatore Lauro - hanno focalizzato criticità e problemi, con situazioni che possono offrire spazi alla criminalità organizzata per ampliare le possibilità di penetrazione e di espansione, di usura e riciclaggio. Ma in questo ambito, se abbiamo le nostre non commendevoli prerogative, siamo peraltro in un'altrettanto discutibile compagnia. Ricordo che la Commissione europea, nel Libro verde attualmente in discussione prima della sua definitiva adozione da parte del Parlamento europeo, ci segnala che dei circa 15.000 siti di scommesse attivi in Europa più dell'85 per cento opera attualmente senza una regolare licenza. Dunque, come ha riconosciuto recentemente il commissario al mercato interno Barnier, la mappatura europea del gioco d'azzardo *on line* è una precondizione decisiva sia ai fini della trasparenza e della regolazione del settore, sia, e soprattutto, per la tutela dei cittadini, specialmente dei minori. Ma c'è da fare molto anche da noi per rafforzare regolazione e controllo, a partire dalla trasformazione di AAMS in agenzia, che è stata annunciata, ma che noi vorremmo vedere più celermente concretizzata, investendo così su una qualificazione delle competenze amministrative, giuridiche, tecnologiche e ispettive di un comparto che è in rapidissima trasformazione; anche perché recenti vicende arrivate agli onori della cronaca nelle passate settimane dicono che bisogna accelerare in questa direzione di irrobustimento dei controlli, della capacità di contrasto e della tempestività di intervento. Faccio un esempio: ho depositato proprio oggi un'interrogazione inerente una società che presenta profili che - cito dalla stampa - potrebbero far venire meno il rapporto fiduciario con ma questo avviene a dieci giorni dall'introduzione del *cash gain* nel sistema di gioco, per cui da luglio sarà possibile puntare fino a 1.000 euro per singole mani mani di gioco e avere poi un rilevante effetto di posta che s'incrementa, e tutto questo attraverso un soggetto che, se non è in rapporto fiduciario con AAMS, genera elementi di opacità in tutto il sistema. Tutti questi elementi inducono alla necessità di ottimizzare e qualificare la capacità di governo di tutto il sistema, ma c'è un ultimo aspetto su cui ci siamo particolarmente impegnati in questa mozione che vorrei evidenziare in questi minuti conclusivi. Viviamo in una fase di criticità per molte famiglie, di difficoltà di potere d'acquisto: ci sono tentazioni molto grandi nel settore del gioco. Il Sottosegretario mi permetterà: ci si è andati un po' di manica larga. Oggi, girando per una città, la presenza di apparecchi da intrattenimento in agenzie, sale bingo, sale giochi, corner, ricevitorie, tabaccherie, bar, ristoranti, edicole, alberghi, stabilimenti balneari qualsiasi esercizio in possesso delle previste licenze, persino dai barbieri, si potranno avere opportunità di gioco. Se poi ci mettiamo tutta la parte del gioco *on line*, si è davvero messi

proliferazione, che abbiamo abbandonato con improvvide misure decise nei decreti dell'anno scorso. L'aspetto che però m'interessa mettere maggiormente in evidenza

entrando dentro una spirale che consegna allo sviluppo delle patologie, della dipendenza da gioco, con tutte le implicazioni drammaticamente negative che possiamo conoscere. proprio perché si prospettano nella manovra addirittura ulteriori aperture con la previsione di ulteriore incremento di gettito, abbiamo bisogno che ci sia da parte dello Stato l'esercizio della responsabilità: governare un sistema, e non disdegnare il fatto che ci possono essere introiti per la collettività e l'erario, ma anche avere attenzione a tutelare i soggetti deboli e sviluppare le azioni di regolazione e trasparenza che aiutino a rafforzare le difese contro un mercato che potrebbe essere eccessivamente invasivo e generare delle conseguenze negative in termini di diffusione di patologie, come hanno già ricordato altri colleghi nei loro interventi, illustrando le diverse mozioni. Per tali ragioni, la nostra mozione si conclude con una sollecitazione, sapendo che il Governo il Governo è impegnato ad emanare una disposizione su questo tema proprio per prevenire e contrastare i fenomeni di ludopatia conseguenti al gioco compulsivo, prevista nella legge di stabilità per l'anno 2011. Sollecitiamo con questa mozione il Governo a concentrarsi sulla necessità di adottare misure finalizzate a regolamentare formalmente e specificamente ogni forma di pubblicità sui giochi d'azzardo, in senso lato e caso per caso, allo scopo di limitare i rischi per il consumatore e in particolare, per i giovani di subire messaggi distorti ed ingannevoli. Basta guardare la televisione per ricevere qualche monito ed esempio di come si sta procedendo inoltre il Governo ad adottare, come si è fatto per il fumo, meccanismi di dissuasione. Ad esempio, sui gratta e vinci e su altre forme di lotterie cartacee ci potrebbero essere

inoltre possibile determinare, soprattutto rispetto al tema dei minori, che è stato richiamato, delle soglie di sbarramento per l'accesso, in modo da evitare che, in particolare tra i minori, vi sia una diffusione impropria di comportamenti e di atteggiamenti che possono generare un sacco di complicanze.

abuso del gioco, per l'attuazione di misure di assistenza e appoggio da parte delle strutture e dei servizi socio-sanitari, per la cura delle forme patologiche e compulsive di dipendenza dal gioco. Chiediamo ancora che sia data attenzione allo sforzo di monitorare in sede comunitaria e di armonizzare una serie di strumentazioni normative di controllo, perché se non si

stanno facendo. Abbiamo apprezzato anche noi le mozioni presentate dagli altri Gruppi: mi pare che ci sia una convergenza, al di là delle sfumature di sensibilità e di impegno. Ci sarebbe la possibilità - credo che ci sia stato anche un impegno del Sottosegretario in questo senso, e io lo caldeggio

che tale industria sviluppi una capacità produttiva di *software*, di occupazione e anche del divertimento, ma in una forma tale da tutelare i più deboli e da evitare che si determinino anche per questa via iniquità e sofferenza sociale.

è di grande rilevanza sociale. Richiamando quanto poc'anzi ha dichiarato il senatore Lauro, consideriamo l'approccio odierno introduttivo di un dibattito più approfondito che vorremmo potesse svilupparsi sul documento che la Commissione antimafia licenzierà nei prossimi giorni. Vi sono alcuni dati che dimostrano l'importanza del tema che stiamo affrontando.

nel 2009 è stata pari a 53,773 miliardi; nel 2010 - il comunicato ufficiale è dei Monopoli di Stato

Nel giro di quattro anni la raccolta da gioco è aumentata del 400 per cento.

ogni italiano, da zero a oltre cento anni, spende nel gioco 2.000 euro ogni anno. C'è un dato che inquieta: i giorni di aumento delle giocate nel corso dell'anno, in particolare del gioco rappresentato dalle macchine elettroniche e dai gratta e vinci, coincidono con i giorni di riscossione delle pensioni. Nei momenti di crisi economica del Paese, la prospettiva della vincita costituisce l'ambizione di una massa enorme di italiani. Il fenomeno così diffuso mette poi in evidenza la parte patologica, ossia l'esistenza

le cronache ci hanno infatti consegnato la tristissima pagina di quei due genitori che, a distanza di pochi giorni, hanno lasciato i loro bambini, di pochi mesi e di pochi anni, chiusi in macchina perché dovevano recarsi a giocare ai videogiochi. Questa è la deviazione pesante, la malattia che sta infettando in profondità il popolo italiano. Noi non possiamo stare a guardare.

che lo Stato è indirizzato a recuperare risorse dal settore dei giochi «i cui proventi netti possono possono ormai continuare a crescere solo grazie a un'espansione esponenziale del volume della raccolta. Il consumo di giochi interessa prevalentemente le fasce sociali più deboli e culturalmente meno attrezzate: la forzatura su tale fonte di entrata non può, dunque, non sollevare qualche fondata perplessità».

i giocatori vincono, anche: quindi una parte della spesa da gioco rientra con le vincite. Senonché, è scientificamente dimostrato che il giocatore che vince rigioca, perché il meccanismo infernale non si ferma mai. Se si vince un euro con un gratta e vinci, si reinveste per acquistare un altro biglietto, se se ne vincono due si comprano due biglietti. Il cittadino perde sempre.

per una grande fetta, a favore di chi in regime di monopolio gestisce il settore, creando enormi bacini di liquidità

si utilizza il canale dell'usura, si sollecita il giocatore, che spesso e tanto frequentemente - sono numeri impressionanti - impegna anche la propria casa o aliena i propri esercizi commerciali. Sono drammi infiniti.

l'economia degli italiani, delle famiglie e dei singoli. Riporto i dati del 27 maggio 2011. Le videolotterie - gli apparecchi da intrattenimento di ultima generazione - installate sono salite a 21.881 e, a regime, le videolotterie, i nuovi strumenti da gioco, arriveranno a 57.000. Oggi esistono 383.008 apparecchi, le *slot machine*, con regolare concessione; tolta una quota che va in magazzino per riparazione, le macchine in esercizio sono 342.311. Non se ne può più. Dovunque c'è offerta da gioco; dovunque si cerca di prendere denaro dalle tasche dei singoli cittadini. Dobbiamo fermare questa deriva, perché quando si infetta un Paese a certi livelli il recupero diventa difficile. E non è soltanto il recupero dalla disperazione: è il recupero da una malattia.

la possibilità di prevedere un trattamento terapeutico. Invece, i primi tagli della sanità riguardano proprio questo settore, in quanto la ludopatia non è ancora considerata considerata una malattia scientificamente accettata e quindi sfugge all'assistenza terapeutica. Ecco, noi offriamo un fianco di grande debolezza. Ma voi vi accorgete di quanta raccolta da gioco avviene via Internet, con piattaforme collocate all'estero, che raccolgono

si vedono continuamente videolotterie; il *videopoker* si trova ovunque. Spesso si tratta di società che operano all'estero e che non versano all'erario neanche un euro perché sfuggono a qualsiasi controllo. Quindi, l'erario subisce anche un danno da questo fenomeno. Si incentiva la malattia, ma a lucrare sono i banditi che utilizzano la malattia per fare soldi. Ecco perché nella nostra mozione sollecitiamo ciò che è stato un punto di approdo della Commissione antimafia, ossia estendere l'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza anche alle piattaforme che operano all'estero, richiedendo quindi l'autorizzazione prevista dal Testo unico di pubblica sicurezza anche per quelle piattaforme. Dato che non si potranno regolarizzare le loro posizioni, ci sarà la possibilità dell'oscuramento dei siti (è strumentale la nostra richiesta

almeno impegnare il Governo ad aiutarci a contrastare questo fenomeno, che sfugge a qualsiasi controllo. Questo è l'inizio di un discorso che noi speriamo di poter svolgere in questa legislatura in maniera

Noi dobbiamo riportare le regole, per difendere il cittadino e per combattere la criminalità organizzata che su questa nuova frontiera ha investito e lucra. Ci deve essere uno sforzo di tutte le forze politiche - e tutte le mozioni vanno in questa direzione direzione - e del Governo, che nell'ultima legge di stabilità ha inserito la necessità di intervenire per contrastare la ludopatia. che, nel momento in cui si individua la necessità di contrastare la malattia da gioco, poi non possa esserci, dopo due commi della legge di stabilità, la previsione di incentivare l'offerta da gioco, autorizzando l'immissione nel mercato

Questa è una malattia sociale pesantissima. Non è qualcosa su cui si possa essere distratti. Quindi, affido alla vostra considerazione e alla considerazione, che penso positiva, del Governo, avendo prima avuto occasione di confrontarci, questa mozione. Ovviamente, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà a favore delle mozioni di tutti gli altri Gruppi.

La mania del gioco è un fenomeno che negli ultimi 15 anni è cresciuto in modo esponenziale, con un incremento del ricavato soprattutto per le casse dello Stato.

*Slot machine*, *videopoker* e *casinò* *on line* sono i nuovi strumenti della mania del gioco, definita tecnicamente ludopatia. La febbre del rischio diventa una vera e propria mania, un'ossessione per il gioco d'azzardo,

La mozione che oggi stiamo discutendo, come credo sia facile capire, tratta una problematica di una complessità e di una gravità veramente estreme. Il problema della dipendenza dai videogiochi sta assumendo negli ultimi tempi, come diciamo da tempo, proporzioni di sempre maggior rilievo. Migliaia di persone finiscono purtroppo sul lastrico per colpa dell'ossessione per le cosiddette macchinette Il gioco d'azzardo è definito una dipendenza, e chiaramente i numeri e la portata di questo fenomeno ci fanno capire che effettivamente stiamo parlando di totale dipendenza. Gli esperti del settore definiscono questa patologia come dipendenza senza droga

L'esplosione del mercato del videogioco è legata a tanti fattori, primi fra tutti la liberalizzazione del mercato e l'ampliamento di modalità di gioco che hanno portato al settore nuovi operatori e soprattutto anche nuova tecnologia. Il fenomeno, lo si evince dai numeri, è complessivamente in crescita e purtroppo interessa soprattutto i giovani. La metà degli studenti italiani ne sono coinvolti con un incremento maggiore tra le ragazze. ragazze. Gratta e vinci, lotterie istantanee, scommesse sportive, lotto e superenalotto sono i giochi in denaro più praticati. I minorenni scolarizzati che scommettono illegalmente sono più di mezzo milione nel nostro Paese.

Molta gente, purtroppo molti giovani, molti adulti, molti anziani ne sono coinvolti. I numeri sono impressionanti e ai numeri leciti e ufficiali, nonostante la liberalizzazione del fenomeno, dobbiamo purtroppo aggiungere tutto il fatturato che proviene dal giro clandestino del gioco sommerso.

La crescita del fenomeno ha naturalmente fatto emergere oggi una versione più evoluta di chi gestisce questi giochi, che vengono definiti cravattari, ovvero coloro che prestano denaro a strozzo. Accade dunque che i cosiddetti prestiti già da qualche tempo sono concessi per finanziare le giocate, un fenomeno che coinvolge direttamente operatori economici, commercianti, piccoli imprenditori; quindi, anche il mondo dell'economia ne è inevitabilmente coinvolto. Si gioca con l'illusione di poter superare le difficoltà finanziarie, a volte cercando di superare anche i problemi della propria azienda.

Occorre però consapevolmente riflettere oggi sull' opportunità di non compiere un passo indietro nel porre veti che oscurino un percorso di trasparenza nell'utilizzo dei videogiochi, in quanto, a volte, il vietare può condurre ad alimentare il gioco d'azzardo non controllato e pertanto alla pericolosa ipotesi del gioco che diventa illecito e quindi subito appannaggio

Le campagne di sensibilizzazione sono sicuramente vincenti; con queste metteremo in evidenza tante problematiche che nascono dal videogioco. Siamo convinti che il Governo si attiverà in questa direzione

Il livello di benessere sociale di un Paese si misura anche con il ruolo che lo Stato svolge per evitare che certi fenomeni assumano la rilevanza di problema. È necessario intervenire

infatti è stato già ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, il gioco d'azzardo patologico è un disturbo del comportamento che, pur rientrando tuttora nella categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle cosiddette dipendenze senza sostanze. Il giocatore patologico, infatti, mostra una crescente dipendenza nei confronti del gioco d'azzardo aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, la somma spesa nel tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco. Con la crescente legalizzazione di giochi d'azzardo aumentano gli individui che entrano in contatto col gioco. La popolazione adulta dei Paesi industrializzati con disturbi da gioco d'azzardo patologico è stimata tra lo 0,5 e il

In Italia la cura dei giocatori patologici è effettuata, anche se in modo ancora non omogeneo, dai servizi di tossicodipendenze delle ASL (i che sono generalmente in grado di fornire informazioni sui centri di cura anche quando non se ne occupano direttamente. Naturalmente, vanno supportati e potenziati, dato che ad oggi,

si potrebbe contrastare il fenomeno e restituire uno stato di benessere psico-fisico alla persona dedita al gioco. Non vanno dimenticate poi, come ricordato dal senatore Vallardi, le campagne di sensibilizzazione, educazione e prevenzione in genere rivolte a tutta la popolazione ma soprattutto ai giovani che a volte, per spirito di emulazione nei confronti dei soggetti adulti, intraprendono una strada non solo dalla quale è difficile uscire, ma che porta con sé la potenziale predisposizione a compiere atti delinquenziali connessi come, ad esempio, rubare per procurarsi denaro con cui giocare. Pertanto, come tutti i fenomeni di dipendenza, è chiaro che la strada da intraprendere è la prevenzione e l'informazione, come è stato fatto con le campagne contro il fumo, soprattutto nei confronti dei più giovani anche nelle scuole,

ho anche riscontrato una sensibilità forse oggi maggiore rispetto all'altro ramo del Parlamento su questi argomenti. E proprio in questa sede, già su altri provvedimenti, avevamo verificato

Partirei da una riflessione ampia. In questi mesi, abbiamo affrontato molto spesso la materia del gioco, cercando di alzare l'asticella

per presidiare, ovviamente, il mercato dei giochi (che, comunque, esiste e che ha una naturale declinazione oggi nel nostro Paese, a prescindere dall'offerta che può essere fatta dall'attività dei Monopoli di Stato, in relazione alle concessioni fino ad oggi date) ma, più in generale, per svolgere un'attività costante per normare alcuni fenomeni che rappresentano oggi una novità significativa e con percorsi di crescita straordinari.

concluso un accordo di cooperazione tra l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e l'autorità francese, l'ARJEL, relativamente al presidio di questo settore, allo scambio di informazioni tra Francia e Italia,

la Francia ha adottato una normativa similare proprio nel marzo 2010 e, grazie a questa attività costante di relazione intercorsa negli ultimi due anni, si è costituito questo accordo che ci consentirà di presidiare in modo più efficace l'attività del gioco lecito, in Italia e in Francia, ma, allo stesso tempo, di perseguire attività illecite con strumenti e informazioni nuove.

in cui credo che il regime concessorio, che rappresenta un elemento di specificità non solo nazionale ma anche internazionale, possa essere considerato e guardato anche dagli altri Paesi come modello di riferimento. É evidente che, nella materia dei controlli, e tratterò soprattutto questo aspetto, molto è stato fatto in questi anni, e molto resta da fare. È giusto però ribadire che i controlli comunque sono stati fatti e che c'è stata, in ogni caso, una determinazione dei compiti assegnati ai Monopoli di Stato dalle norme e dalle direttive dell'autorità politica. Insieme alle forze dell'ordine è stata svolta un'attività che io ritengo di assoluta importanza. In particolar modo, noi riteniamo che la legge di stabilità per il 2011 abbia rappresentato, e rappresenti oggi, un punto di riferimento importante importante per le iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi. L'intervento ha operato su diversi profili. Innanzitutto, siamo intervenuti sul piano della prevenzione; l'articolo 1, comma 77 e seguenti della di stabilità ha previsto l'introduzione di più stringenti requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento in concessione (questo è stato un elemento assolutamente nuovo rispetto al passato) al passato) in tutti i settori di gioco pubblico, sia in ordine alla trasparenza degli assetti proprietari delle società concessionarie (tema che è in qualche misura ricorrente anche all'interno delle mozioni), sia con riferimento alla solidità tecnico-organizzativa e patrimoniale delle stesse. La nuova disciplina concessoria, attraverso lo strumento di appositi atti aggiuntivi, sarà applicata anche alle concessioni vigenti entro il corrente mese di giugno, in linea con la tempistica prevista dalla legge di stabilità. Sotto il profilo dei controlli, ricordo che il comma 80 del predetto articolo 1 ha introdotto specifici ulteriori poteri di controllo ed ispettivi affidati ai Monopoli di Stato in caso di concessione e l'introduzione di ulteriori sanzioni per l'inadempimento degli obblighi convenzionali. Attiene sempre al rafforzamento degli strumenti di contrasto al gioco irregolare e alle infiltrazioni criminali, in particolare nel settore specifico delle *newslot*, sia la previsione del censimento degli apparecchi e delle relative ubicazioni che l'istituzione dell'elenco dei soggetti che operano a vario titolo nella filiera, per i quali tutti sono previsti specifici requisiti di carattere soggettivo. Sono due elementi che abbiamo considerato fondamentali, fondamentali, per riconoscere, attraverso un albo concessorio vero e proprio - in cui ci sono anche le caratteristiche dei cosiddetti gestori e si va a ricomprendere un innalzamento di trasparenza, e ovviamente di presidio della legalità all'interno di tutta la filiera - non solo il concessionario con questi nuovi presìdi di carattere normativo, ma anche, ovviamente, i gestori e gli operatori: tema che fino a qualche mese fa era comunque una questione che non veniva mai trattata e presentava anche un *vulnus* normativo. La stessa legge di stabilità per il 2011 ha previsto, inoltre, un piano straordinario di controlli, che stiamo espletando, con riferimento in particolare ai settori del gioco *on line*, delle scommesse e degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento. In particolare, per quanto attiene al gioco *on line*, nel corso del corrente anno, a seguito della raggiunta operatività del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15-*ter* del decreto legge 1° luglio di cui fanno parte rappresentanti dei Monopoli di Stati, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (comitato voluto espressamente dal Governo e dai Monopoli di Stato), sono già state pianificate alcune operazioni di contrasto all'illegalità (di cui alcune svolte proprio nei giorni scorsi), sull'intero territorio nazionale, con la partecipazione sinergica di tutte le forze di polizia. La prima di tali operazioni, relativa al settore delle *newslot*, ha già avuto luogo nella prima settimana dello scorso mese di maggio ed è stata indirizzata principalmente a contrastare l'offerta di gioco a minori di anni 18 e ha interessato, nell'arco di 48 ore, migliaia di esercizi. Nel settore del gioco *on line*, ed in particolare dell'offerta da parte di siti non autorizzati, l'attività di contrasto, che si giova della fattiva collaborazione della Polizia postale, ha portato, dall'inizio del corrente anno ad oggi, all'inibizione di 378 siti che operavano fuori della legge. Vorrei anche ricordare, colleghi, che voi avete trattato giustamente l'importanza della questione del gioco *on line* e dei presidi da guadagnare. Mi permetto di sottolineare che, quando noi abbiamo in qualche misura proposto la norma all'attenzione del Parlamento, c'erano delle versioni più stringenti: avevamo ipotizzato di costituire un vero e proprio portale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; avevamo immaginato anche azioni che fossero ancora più chiare dal punto di vista della comunicazione su ciò che doveva essere considerato gioco e raccolta del gioco a distanza lecito rispetto al al gioco illecito. È evidente che la logica del confronto parlamentare ha portato in qualche misura ad abbassare un po' il profilo dell'intervento che era stato immaginato dal Governo, ma questo lo dico proprio perché, a distanza di tempo, la sensibilità che oggi raccolgo in Parlamento - e ne siamo felici - punta ad alzare il presidio della legalità. E il Governo non si sottrae: trarrà spunto da queste mozioni per rafforzare le iniziative che svolgeremo nei prossimi tempi, anche dal punto di vista normativo. La Guardia di finanza, competente all'accertamento delle violazioni all'obbligo di oscuramento dei siti *web* illegali, provvede a monitorare i siti Internet per i quali i Monopoli di Stato hanno emesso il provvedimento di inibizione, interessando successivamente i reparti territoriali competenti in relazione alla sede del *provider*, per verificare che la connessione ai siti irregolari sia stata effettivamente reindirizzata verso la pagina *web* predisposta dai Monopoli di Stato e, in caso negativo, la contestazione ovviamente della prevista sanzione amministrativa che va da gennaio 2009 a maggio 2011 i reparti del Corpo hanno effettuato complessivamente 15.389 interventi, all'esito dei quali sono stati verbalizzati 20.157 soggetti, sequestrati 10.000 apparecchi e 3.467 punti clandestini di raccolta scommesse. Sul piano operativo, l'azione del Corpo si è caratterizzata per un approccio di carattere trasversale volto a colpire tutte le manifestazioni di illegalità economico-finanziaria connessi ai fenomeni di abusivismo e clandestinità scoperti: dalla verifica del possesso di licenze, autorizzazioni e concessioni di legge alla corrispondenza delle caratteristiche dei giochi ai requisiti previsti dalla norma, dal corretto ed effettivo pagamento dei tributi al contrasto degli interessi e delle ingerenze della criminalità nel settore. Per finalità di contrasto al riciclaggio perpetrato questo specifico comparto i reparti di Guardia di finanza effettuano, unitamente alle indagini di polizia giudiziaria, lo sviluppo investigativo delle segnalazioni per operazioni sospette generate dal sistema finanziario svolgono ispezioni presso gli intermediari, i professionisti e altri operatori non finanziari per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo. serve per dire quanta evoluzione c'è stata sul versante dei controlli. L'altro aspetto fondamentale è il percorso di formazione costante delle forze dell'ordine su questa tematica così complessa. Al fine di evitare che il settore delle scommesse si trasformi in uno strumento per il riciclaggio di denaro sporco, il decreto legislativo n. 231 del 2007, successivamente integrato dal decreto legislativo n. 151 del 2009, ha introdotto specifici obblighi in capo agli operatori che esercitano, sia in sede fissa che con la modalità *online*, l'attività di offerta di giochi. Siamo in fase di emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Anche se in ritardo, siamo alla conclusione dell'*iter*, abbastanza complicato dal punto di vista tecnico.

e sono state riscontrate irregolarità a vario titolo in relazione a 12.717 apparecchi, che rappresentano il 13 per cento del totale degli apparecchi controllati. Potrei andare avanti, perché sono molti i dati,

legge-quadro complessiva del settore del gioco, portando qualche ulteriore elemento di innovazione che potrà raccogliere alcuni stimoli posti dalle mozioni e riuscendo anche a innalzare ulteriormente il livello di attenzione su alcune problematiche connesse alla diffusione del gioco, anche di quello lecito. Sappiamo che alcuni problemi ci sono

Nell'ambito del nuovo Piano sanitario nazionale 2011-2013, in corso di adozione, è previsto uno specifico piano di azioni mirato all'individuazione degli interventi prioritari da porre in essere in varie aree di bisogno, tra cui i disturbi psichici correlati alle dipendenze patologiche e i comportamenti da abuso. Aggiungo inoltre che il Ministero della salute sta predisponendo, con il Ministero dell'economia e delle finanze, di Stato e il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio, il decreto previsto all'articolo 1, comma 70, della legge di stabilità per il 2011. Tale decreto, nel rispetto della norma di rango primario citata, reca le linee di azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero dei fenomeni di ludopatia conseguenti al gioco compulsivo. Ciò premesso, e condividendo in pieno la rilevanza anche sociale della problematica posta, in merito all'utilizzo obbligatorio di una tessera elettronica, ci sono alcuni problemi che stiamo cercando di superare. In sintesi, si sta dando attuazione alla norma prevista dalla legge di stabilità, ben sapendo che già altri strumenti sono stati attivati, come un numero verde specifico cui risponde oggi un centralino che dà risposte e immediate indicazioni verso la rete esistente, non ancora organica, ma che rappresenta un passo in avanti.

l'inizio del sesto capoverso

il Gruppo di Coesione Nazionale-Io Sud non ha presentato una sua mozione, anche se ci siamo interessati in altri momenti di questo problema che - come è stato rilevato da tanti colleghi che sono pregevolmente intervenuti intervenuti - è ormai veramente da intendersi come un serissimo problema di carattere sociale. Vediamo che, soprattutto nelle zone più povere del nostro Paese, si fa affidamento sulla dea bendata per tentare di migliorare le sorti personali o, addirittura, della propria famiglia, investendo purtroppo nel gioco - non voglio parlare del gioco d'azzardo perché credo che il gioco in sé rappresenti comunque e sempre una sfida e un azzardo

D'altra parte, il fenomeno sociale è rapportato anche con le cifre, più volte ricordate, degli introiti che derivano dal gioco, ci dicono quanto forte e importante sia questo fenomeno. In questo senso abbiamo molto apprezzato l'intervento del Sottosegretario, che si è mostrato forse insolitamente -

c'è indubbiamente una grande attenzione al fenomeno, soprattutto nei suoi due aspetti fondamentali. Il primo è quello della repressione del fenomeno, con tutti quanti i mezzi di controllo che si possono porre

che è molto più delicato e anche più difficile da aggredire, soprattutto in queste nostre città che - come sa bene chi ha fatto l'amministratore - sono diventate una sorta di casinò diffuso.

sono suggestivi, non soltanto per la denominazione che hanno, ma perché lo sono nei riguardi della gente che si sente particolarmente attratta dal gioco.

che riguarda una sorta di federalismo rispetto agli introiti che provengono dal gioco. Stiamo parlando da tanto tempo di federalismo fiscale, ma è come se gli introiti che provengono dal gioco gioco - mi riferisco ovviamente al gioco lecito - debbano essere semplicemente appannaggio del Governo centrale: così non è

Recepisco le richieste del sottosegretario Giorgetti in ordine alle modifiche della mozione a mia prima firma; apprezzo notevolmente, come ho già detto, il lavoro svolto da tutti i colleghi con le mozioni e nella discussione: si tratta di una pagina importante dei lavori di questa Sottosegretario Giorgetti, abbiamo colto il suo particolare apprezzamento per questo ramo del Parlamento, che ha manifestato una spiccata sensibilità al problema. È ovvio che ci interessano i cittadini e ci interessa contrastare la criminalità organizzata. Voglio fornire solo un dato. Quando le macchine non funzionano o sono prive di concessione è previsto dalla legge l'immagazzinamento, ossia, le macchine vengono messe in magazzino; in un accertamento fatto alcuni anni fa è risultato che un solo concessionario, in uno stesso giorno, aveva messo in magazzino

e avendo apprezzato anche gli impegni assunti dal sottosegretario Giorgetti, noi della Commissione antimafia continuiamo il nostro lavoro, siamo sicuri di incontrarci;

il problema che mi sembra sia emerso concerne il rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini più fragili. Bisognerebbe riuscire a trovare un tratto di coerenza, perché dal 2002 al 2007 sono cambiati i metri quadri entro cui si possono collocare le macchine.

Quella che c'è sotto casa mia restituisce uno straordinario spaccato di umanità, perché vi entrano tutti i poveri diavoli che tutti noi del quartiere sappiamo non avere di cosa vivere. Può anche darsi che valgano sicuramente i richiami alla responsabilità (bevi con misura,

non per eliminare libertà che non vanno eliminate, ma per capire che in un momento difficile forse anche dare un segnale eticamente certo ("basta, non istalliamone più!") potrebbe essere una speranza alla quale aggrapparsi seriamente.

precipitano in un altro baratro. Oggi è stato citato tante volte Gibran, lasciatemi citare in conclusione la solita canzonetta: non c'è vuoto, non c'é vuoto davvero che possa in qualche modo essere riempito, perché la vita non è un gioco.

Si parla di macchinette che arrivano a distribuire vincite fino a 5000 euro, cifre importantissime, con *jackpot* (che non so nemmeno come funzionino) che portano a vincite complessive di 100.000 euro.

coperti da *privacy*, un cittadino non possa spendere nel gioco più di quanto porta a casa la famiglia (per evitare che famiglia e figli restino privi di sostegno economico, e io aggiungo alimentare) è già un grande passo. È questo che chiediamo al Governo e lo ringraziamo per aver accettato la nostra proposta. onorevoli colleghi, c'è un dato sopra tutti che ci impone di assumere da oggi impegni chiari e urgenti e l'individuazione di un percorso serio e responsabile sul fenomeno, qual è quello del gioco d'azzardo, che negli ultimi anni ha assunto una dimensione così rilevante per portata ed intensità. Il dato cui mi riferisco è la continua e crescente diffusione del gioco e il conseguente rischio di dipendenza tra i minori, ragazzini nella fascia di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Parto da questo dato (ce ne sarebbero molti altri) perché credo sia emblematico della gravità del tema che stiamo affrontando. Le domande che quel dato suscita ci interrogano sulla rilevanza etica e sulle conseguenze del gioco d'azzardo; ci chiedono di intervenire con la massima urgenza, pena una colpevole sottovalutazione di un allarme sociale tanto più problematico se coinvolge in parte anche i minori; ci sollecitano a non abdicare al ruolo di regolamentazione che lo Stato deve assumere in un settore che tocca i principi del vivere civile. Il fenomeno del gioco d'azzardo, infatti, ha connessioni economiche, sociali, sanitarie, e più in generale culturali, che si intrecciano in una complessità che richiama appunto i fondamentali del nostro vivere comune. Nel 1990 il settore muoveva circa 5 miliardi di euro, nel 2010 ne ha mossi più di 60: il 1.100 per e, come ha detto il senatore Barbolini, già nel primo semestre di quest'anno siamo ad un'ulteriore 20 per cento in più, con un *boom* impressionante, soprattutto nell'ultimo decennio, che non accenna a diminuire e che si insinua profondamente nella parte più debole e fragile della popolazione: giovani, disoccupati, anziani, donne, e proprio nei momenti di maggior crisi economica. L'illusione della vincita facile, la speranza della fortuna a portata di mano, la possibilità di un eventuale riscatto sociale alimentano ed ammorbano questo fenomeno. Negli anni si è ampliata l'offerta istituzionale, con l'introduzione di sempre nuove tipologie di gioco. Si sono ampliate le occasioni spazio-temporali, con un infittirsi della rete dei punti vendita. Non vi è luogo fisico oggi dove non si possa giocare: ogni spazio della quotidianità è stato occupato; la tecnologia informatica ha espanso ulteriormente, in modo massiccio, la capillarità della rete e la facilità del suo utilizzo. I termini orari di accettazione delle giocate si sono prolungati a dismisura; si è ampliata inoltre quella pubblicità positiva che i mezzi di informazione avevano contribuito a diffondere, tramutando quel disvalore sociale del ricorso al gioco d'azzardo, che ha caratterizzato in alcuni momenti la storia del nostro Paese, in un atteggiamento favorevolmente incentivato. È divenuta, cioè, una pratica socialmente accettata. Tutto ciò rischia di avere effetti perversi anche per quanto riguarda l'offerta pubblica di gioco e rischia di ingigantire le conseguenze negative di un'abitudine ormai molto estesa di gioco compulsivo e poco responsabile. Tutto ciò, inoltre, come è stato ben detto anche da chi mi ha preceduto, rischia di rendere sempre più debole la differenza tra lecito ed illecito. Non da ultimo, occorre evidenziare risvolti dannosi e degenerativi, spesso visibili nel lungo periodo, che la pratica dell'azzardo può produrre. Ludopatia, ripercussioni sui rapporti familiari e interpersonali, indebitamento e ricorso a prestiti usurari. Sono costi troppo elevati per la nostra società per lasciarci indifferenti. Per questo credo che non ci si debba limitare al contrasto del gioco illegale, terreno fertilissimo per la malavita organizzata e che comunque non sembra negli anni avere un'inversione di tendenza, pur con la liberalizzazione del gioco d'azzardo istituzionale, con le domande che all'inizio ci poneva il senatore Lauro. Pensiamo da ultimo ai fatti recenti legati al calcio-scommesse con le indagini in corso proprio nella mia città, a Cremona. Ma occorre poi una strategia di prevenzione, informazione, educazione, cultura e presidio di legalità, assistenza e cura per le forme patologiche, come hanno ben espresso sia il senatore Barbolini che la senatrice Biondelli. Abbiamo più volte in questi anni sollevato questi temi, evidenziando come il principio di cautela nella gestione del comparto dei giochi pubblici non costituisca una forma di proibizionismo, trattandosi invece di cautela nella gestione; questo principio dovrebbe essere prevalente rispetto alle esigenze di cassa volta a incrementare le entrate pubbliche. In questi anni, mentre chiedevamo una riforma organica del sistema e proprio mentre la crisi economica induceva ad un ricorso massiccio alla pratica del gioco d'azzardo, determinando così anche una sorta di ulteriore aumento di tassa sui poveri, il Governo è intervenuto più volte in modo invece disorganico, inserendo vari commi nei diversi decreti economici ma mai affrontando la questione nel suo insieme. Con il sottosegretario Giorgetti abbiamo avuto modo di confrontarci in Commissione finanze parecchie volte. Lo ringrazio anche oggi per la competenza, puntualità e completezza nei dati; però, da tempo stiamo chiedendo quella riforma strutturale di cui tutti oggi abbiamo sottolineato l'urgenza. C'è un punto in comune in tutte le mozioni presentate ed è quello di impegnare il Governo in interventi che favoriscano la diffusione di una filosofia del gioco responsabile. Per fare ciò, serve il coordinamento tra i vari Ministeri coinvolti, tra i soggetti chiamati a gestire il settore dei giochi e - noi aggiungiamo con la nostra mozione - il coordinamento a livello europeo. Noi voteremo a favore di tutte le mozioni, però sostenendo quanto detto dal senatore Lauro: si deve trattare di un dibattito introduttivo, soprattutto in vista della legge quadro complessiva

Signor Presidente, sono stati evocati numerosi temi. la famosa frase di Platone secondo cui la fortuna non è altro che la virtù applicata alla vita concreta non ci faccia desistere da questa

anche se, in una società complessa come la nostra, per scomodare Max Weber e lo spirito del capitalismo, la fortuna non si cerchi attraverso il lavoro e l'impresa e non piuttosto con i gratta e vinci e le giocate con

Teniamo conto che nel nostro ordinamento, sin dalla prima legge di pubblica sicurezza del 1865 (allegato B), si discusse a lungo su come contrastare il gioco d'azzardo per sostenere i valori fondamentali della nostra Nazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalla Commissione antimafia potremo ricavare un'ottima sinergia di interventi legislativi, valutando il documento che sta per essere approvato e che traccia traccia le linee essenziali di una iniziativa che potrebbe dare maggiore efficacia e coerenza al nostro sistema normativo ed istituzionale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per farla breve, l'intervento normativo che ci si aspetta sulla materia penso debba tutelare in prima analisi i minori, coprire tutta la parte sulla pubblicità ingannevole, porre particolare attenzione alle scommesse e al registro degli scommettitori, in relazione ai reati di riciclaggio e di usura. Ma va fatta molta chiarezza anche sull'applicazione della direttiva Bolkestein, sulla possibilità di aprire nel nostro Paese delle agenzie di gioco per conto di imprese che che hanno sede nei Paesi dell'Unione europea e che richiedono un intervento reinterpretativo del principio comunitario della libera circolazione dei servizi:

deve essere normata secondo il dibattito che si è svolto in quest'Aula, e credo che potremo farlo mettendo a confronto la libertà dei cittadini di utilizzare uno strumento di svago, quale appunto il gioco, senza compromettere però i livelli di sicurezza e di libertà del nostro Paese, che sono gravemente inquinati anche dalla criminalità, individuale e organizzata. Certamente, far emergere attraverso sistemi legali il gioco che si svolge serve anche a contrastare i sistemi di copertura illegale e di intervento della criminalità. Tutto ciò deve essere fatto con un complesso di principi e diritti fondamentali che credo il Parlamento possa avere la possibilità di delineare in una riforma organica, che naturalmente richiami i principi qui evocati e che si radicano nel codice penale e nella legge di pubblica sicurezza del 1931 e in altre leggi speciali.

Il Governo ha espresso parere favorevole su tutte le mozioni presentate, condizionandolo ad alcune riformulazioni che sono state accettate dai rispettivi proponenti. Prima di passare alla

Come è stato già anticipato ai Gruppi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, già previsto per le ore 16 di domani, è stato anticipato alle ore 12, con trasmissione diretta televisiva.

intervenire a quanto sta avvenendo e potrebbe avvenire a seguito della posizione assunta dall'Autorità per le garanzie Immaginate che un giorno intere sezioni della vostra biblioteca vengano rese inaccessibili. Non vi verrà mai detto quali specifici libri e per quali ragioni sono stati rimossi, ma troverete solo un cartello che vi informa che qualcuno da qualche parte e per qualche ragione ha segnalato che i libri di quella sezione violano i diritti di qualcun'altro. Immaginate che anche dagli scaffali accessibili della biblioteca qualcuno rimuova costantemente libri senza che voi o gli altri utenti della biblioteca sappiate quali volumi sono stati rimossi e senza che vi sia data la possibilità di valutare la rimozione di tali libri. Voi forse credete che questo non possa accadere in una democrazia, ma se il diritto d'autore non sarà regolamentato in modo da garantire che anche nella sfera digitale ci sia il giusto equilibrio tra i diversi interessi presenti nella società, da strumento di emancipazione dei produttori dei contenuti esso diverrà inevitabilmente un sistema di controllo e di censura pervasivo. Quanto vuole fare l'Autorità di garanzia per le comunicazioni è in spregio di qualsiasi normativa del nostro Paese. Il diritto d'autore può e deve essere regolato e deve essere regolato dal Parlamento, non può essere regolato da delibere dell'Agcom. Questo è un tentativo che il Parlamento deve sventare e sono lieto che sia proprio

il rispetto della separatezza tra i poteri dello Stato, evitando che l'Agcom prenda provvedimenti che sanno di censura, di bavaglio e che la cultura italiana venga, di fatto, messa sotto chiavistello.*(Applausi

La Presidenza ha comunicato all'Assemblea che, per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio presentata dal Governo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 40, nonché l'articolo 44 del disegno di legge n. 2243, sarebbero andate a costituire un disegno di legge autonomo che il nuovo disegno di legge sarà nuovamente assegnato alla 1a Commissione. Per effetto di questo meccanismo, la Commissione affari costituzionali si troverà a riesaminare daccapo 43 dei 44 articoli che essa ha già esaminato per circa 12 mesi (dal 23 giugno 2010 al 7 giugno 2011), in questo esame potrà accadere che vengano inutilmente ripetute sedute, audizioni, lavoro istruttorio e procedure emendative. In pratica, dovranno essere rivotati i medesimi articoli e la Commissione dovrà nuovamente pronunciarsi sia sul testo che sugli emendamenti. Si tratta, a nostro avviso, di un rovesciamento della logica e dello stesso spirito del Regolamento. Secondo noi, sarebbe stato assai più opportuno stralciare il solo articolo 43, assicurando un *iter* velocissimo in Commissione e in Aula per l'approvazione e, quindi, sopprimere gli articoli rifluiti anche nel decreto sviluppo. Lo avevamo detto, in parte, in discussione generale, ma la scelta è stata diversa. A questo punto, poiché l'Assemblea e la Presidenza hanno assunto le proprie decisioni, chiediamo che la questione sia trasferita nella sede propria. Lo stralcio, secondo l'articolo 101 del Regolamento, può riguardare singoli articoli o singole disposizioni di un provvedimento per la loro autonoma rilevanza. Nel caso in esame, invece, lo stralcio ha riguardato la quasi totalità del testo, determinando una sua incongrua duplicazione. Chiediamo, allora, che la Giunta per il Regolamento sia investita della seguente questione: è ammissibile lo strumento dello stralcio se esso coinvolge la quasi totalità di un provvedimento vanificando, in questo modo, l'esame già svolto in sede referente?